i Gruppi parlamentari hanno proceduto alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, la cui composizione sarà pubblicata nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016***

Voglio iniziare questa relazione ringraziando, innanzitutto, gli Uffici della Commissione speciale, che hanno fatto un lavoro incredibile, ma anche tutte le componenti politiche dell'arco parlamentare per la disponibilità, la competenza e la voglia di risolvere i problemi dei cittadini, ai quali va data una risposta per cominciare ad intravedere una luce in fondo ad un tunnel: non riusciremo a dare quella luce, ma riusciremo quanto meno a fargliela intravedere. Credo che il modo in cui abbiamo lavorato in Commissione speciale, tutti assieme, sia un esempio di come su alcuni temi la politica possa veramente unirsi per dare le risposte che i cittadini aspettano da tempo.

Un vecchio adagio dice che il meglio è nemico del bene. Credo che però, purtroppo, per chi fa politica questo porti un po' di frustrazione, perché cercare il meglio non può esimerci dal fare bene le cose.

Venendo quindi al merito del provvedimento nel testo assegnato alla Commissione speciale del Senato, esso disciplina la proroga e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone RAI e la sospensione del pagamento delle utenze nei confronti delle popolazioni del Centro-Italia colpite dal sisma verificatosi a decorrere dal 24 agosto 2016. Sottolineo «a decorrere» perché uno dei problemi è che dal 24 agosto 2016 non c'è stato un giorno in cui il terremoto non si è fatto sentire in quelle zone.

Nello specifico, il primo comma dell'articolo 1, alla lettera *a)*, apporta modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, disponendo che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché degli esercenti di attività agricole, decorre dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo, invece delle 24 24 attualmente previste. Si aggiunge, altresì, la previsione in base alla quale l'insufficiente e tardivo omesso pagamento di una o più rate comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati, nonché delle relative sanzioni. Si dispone inoltre che in caso di ravvedimento del contribuente non venga eseguita l'iscrizione a ruolo. La lettera *b)* del comma 1 prevede inoltre la proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione, posticipando la data d'inizio del rimborso dal mese di maggio 2018 al mese di gennaio 2019, prevedendo al contempo la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione dagli attuali ventiquattro a sessanta mesi. Il comma 2 proroga dal primo gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, ossia gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS. Le disposizioni contenute nei commi da 3 a 5 dispongono la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni e di interessi, dal primo gennaio 2021. dal primo gennaio 2021. In particolare, l'ambito oggettivo per tale sospensione interessa complessivamente 138 Comuni terremotati, così come individuati dalla legislazione vigente. La norma in esame prevede poi il versamento delle somme oggetto di temporanea sospensione mediante una rateizzazione delle seguenti caratteristiche: fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, mancata applicazione di sanzioni e interessi, decorrenza dei versamenti dal primo gennaio 2021. Anche in questo caso, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si prevede l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati, nonché, in tal caso, delle relative sanzioni e interessi, prevedendosi che la relativa cartella sia notificata, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateizzazione. L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento. Il comma 6 modifica l'articolo 2-*bis*, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, intervenendo sulla sospensione dei pagamenti delle fatture e delle utenze relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia. In particolare viene stabilito che la sospensione sia differita fino al primo gennaio 2019 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. percorsi contenuti nel decreto-legge, che nasce come proroga di adempimenti fiscali e tributari. Vorrei fornire un quadro sintetico dei numeri riferiti alla gestione dell'emergenza forniti dal capo del Dipartimento della Protezione civile, dottor Borrelli, e dal commissario straordinario

Per quanto riguarda le forme di assistenza alla popolazione, il Capo della Protezione civile, in audizione presso la Commissione speciale, ha riferito che all'indomani del 30 ottobre 2016, il numero delle persone che non hanno potuto far rientro nella propria casa è aumentato in modo considerevole; si è passati dai 4.800 assistiti di inizio settembre, a più di 30.000 persone assistite nella prima settimana di novembre, fino ad arrivare alla data odierna a complessive 50.157 persone, di cui 38.668 beneficiari del contributo per autonoma sistemazione (CAS), 7.125 nelle soluzioni abitative di emergenza (SAE), 2.341 in alberghi, 781 nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE), 722 nei moduli *container* e nei *camper* forniti dalla Protezione civile, nonché 520 in altre strutture. I dati che ho citato danno la dimensione della tragedia che queste zone hanno dovuto subire e soprattutto la prosecuzione nel tempo di eventi sismici che hanno causato danni su danni a edifici che già avevano subito la prima scossa. Vorrei inoltre ricordare, come riportato dalla relazione sul sisma del Centro Italia 2016-2017 del Commissario straordinario del Governo, che gli eventi sismici hanno interessato un territorio di quasi 8.000 chilometri quadrati, di cui 2.000 chilometri quadrati inseriti in aree protette o parchi naturali, ed abitato da circa 600.000 persone. Gli edifici esistenti nel territorio delle quattro Regioni sono 185.541, di cui 162.991

Mi soffermo, infine, sui dati relativi ai controlli effettuati sul patrimonio edilizio interessato dagli eventi sismici, evidenziando che si è proceduto ad effettuare oltre 250.000 controlli sulla stabilità degli edifici: 4.600 sugli edifici pubblici, 5.800 sulle chiese e sui beni culturali e la restante parte sul patrimonio edilizio privato. Sono stati accreditati, per il censimento dei danni, oltre 6.500 tecnici, a cui va il mio personale ringraziamento e credo quello di tutta l'Assemblea. I dati numerici poc'anzi riportati mostrano chiaramente come fosse imprescindibile, nel corso dell'esame del provvedimento, procedere ad un'analisi che andasse anche oltre gli ambiti di intervento del decreto-legge, così come adottato del precedente Governo, tenuto conto che, oltre alla questione della sospensione dei versamenti tributari e contributivi, diverse sono le questioni legate alla

di creare aree attrezzate per i proprietari di seconde case per un periodo coincidente con il completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari, di prorogare le scadenze di sospensione dei mutui, prorogare le misure di sostegno al reddito - la cosiddetta cassa in deroga - di esentare le imprese dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per la ricostruzione, almeno nei centri storici e nelle zone rosse, di finanziare gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e igienico-sanitaria, nonché gli interventi di adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, accelerare le procedure per la ricostruzione leggera. La fase di ricostruzione post-sisma risulta essere rallentata non solo dal protrarsi delle scosse, ma anche da lievi difformità urbanistiche ed edilizie sugli immobili tali da impedire il prosieguo del procedimento di concessione dei contributi. Su questo

da parte del tecnico e quindi l'accesso al contributo. Ritengo che uno sforzo in questo senso debba essere fatto e che possa provare a farlo anche l'Assemblea

per cercare di capire se sarà possibile intervenire in modo sensato e concreto sul problema già in quest'Aula. Approfitto per ringraziare anche la fortuna, che ha fatto sì che all'interno della Commissione speciale ci fossero dei sindaci e degli amministratori locali, che vivono sulla loro pelle, ogni giorno, queste tematiche e questi problemi: loro contributo è stato fondamentale per il lavoro della Commissione. e di prevedere la compatibilità tra la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (il cosiddetto sisma *bonus*) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici. È stato chiesto di accelerare il rilancio del tessuto produttivo delle aree colpite duramente dal sisma, sostenendo gli investimenti produttivi, che permettono anche alle piccole imprese di accedere ai benefici previsti dalla normativa. Nel corso del costruttivo dibattito tra i diversi Gruppi parlamentari in Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti, che in buona parte hanno ripreso le istanze sollevate dai vari soggetti ascoltati nel corso delle audizioni. Sono stati approvati - cito qualche dato - 42 emendamenti in totale, di cui sei di *drafting* e sei identici: quindi sono 30 le tematiche che abbiamo affrontato, credo quasi tutte con un voto molto ampio, se non unanime.

una proposta che ovviamente potrà essere rivista in seguito, per prorogare ulteriormente questo termine con la legge di bilancio che verrà fatta da questo Governo, che potrà allocare anche maggiori risorse sulla questione del terremoto, come

è andato a buon fine. Ci sono dei temi che non siamo riusciti a toccare e dei problemi che non siamo riusciti a risolvere.

macerie: le macerie di molti edifici crollati devono essere portate in discarica, ma forse vi sono delle soluzioni alternative per recuperare quelle pietre che sono così importanti dal punto di vista urbanistico e ambientale per quel territorio. Dovrà essere fatta una riflessione urbanistica sulla ricostruzione ampia. Questo tema mette in evidenza la necessità generale per il Paese di rivedere le proprie norme in materia: la legge urbanistica del nostro Paese ha

Tornando, quindi, ai temi toccati in Commissione speciale, che hanno visto poi approvati degli emendamenti e ribadita la proroga dello stato di emergenza, ci sono le disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case. Abbiamo voluto affrontare un tema molto sentito: ampie parti del territorio colpito dal sisma sono composte da edifici utilizzati da famiglie che abitano in un'altra zona del Paese, ma che utilizzavano quegli edifici come seconde case, non tanto per le vacanze, quanto proprio per un radicamento alle proprie origini, che è fondamentale portare avanti. Abbiamo inteso, quindi, proporre la creazione di alcune aree attrezzate per *camper*, per dare la per dare la possibilità a queste famiglie di recarsi in quelle aree e continuare a sentire quel legame forte con le proprie origini, sebbene la loro casa sia stata distrutta. Abbiamo voluto inserire tra i contributi i costi per gli adeguamenti antincendio e per il superamento delle barriere architettoniche. Abbiamo ribadito che, all'interno della richiesta di contributo nel quadro economico, sono compresi anche gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico: si tratta di un costo molto spesso ingente, soprattutto per cantieri che dovranno durare molti anni. Abbiamo disposto una norma che innalza la soglia SOA delle imprese per la ricostruzione tramite appalti privati. un emendamento che prevede una richiesta, tramite legge, al Commissario, che dovrà far fronte a un tema molto sentito e che abbiamo sentito spesso citato nelle audizioni: la chiarezza normativa. La struttura commissariale ha emanato, credo, 59 ordinanze, alcune delle quali ancora in sospensione, su un impianto normativo corposo, ritoccato moltissime volte dal Parlamento, giustamente, perché le esigenze cambiavano nel tempo e c'era bisogno di adeguare gli strumenti normativi. Questo fa sì che oggi un tecnico che debba redigere la pratica per la richiesta del contributo non ha un unico testo su cui lavorare, ma ha di fronte una normativa frastagliata. Abbiamo chiesto quindi che ci sia una linea guida interpretativa unica, in modo da agevolare il lavoro dei tecnici. Abbiamo approvato un emendamento per la proroga dei mutui dei Comuni e delle indennità a favore dei sindaci. Abbiamo approvato alcune norme di semplificazione normativa. Abbiamo approvato proroghe per la sospensione di mutui privati e per le imprese fino al 2020-2021.

di procedere al raggiungimento degli obiettivi sulla raccolta differenziata, quindi era giusto dare un segnale in questo senso. Abbiamo altresì pensato alle esenzioni nella zona rossa per le utenze e affrontato il tema dei condoni pendenti, che non hanno ancora visto il rilascio di certificati di abitabilità e agibilità per carenza documentale e che tengono quindi appese le domande di contributo. In questo senso abbiamo voluto unire il procedimento di accesso al contributo, quindi la progettualità dell'edificio, alla pratica di condono esistente. Abbiamo voluto sanare una situazione che si è creata in diverse parti del territorio, cioè quella di proprietari di case distrutte o gravemente danneggiate che hanno voluto costruire, in modo anche estemporaneo, una piccola costruzione abitativa di fianco alla propria casa, nel proprio terreno di pertinenza, per restare vicino alla alla propria *domus*, quindi alla propria terra. Le situazioni che presentavano delle difformità sono viste ovviamente come emergenziali e andranno demolite al temine dell'emergenza, quindi al rilascio del certificato di agibilità dell'edificio principale; non potevamo certo pensare che queste persone, che hanno fatto uno sforzo per restare su quelle terre, proprio per dare un segnale anche di vicinanza, venissero colpite dalla procura che stava indagando rispetto a eventuali reati. la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per tutto il 2018. Infine, passando agli ultimi due temi, per le imprese con più di 400 dipendenti è stata proposta la cassa integrazione in deroga per i primi sei mesi del 2019.

Ringrazio i proponenti dell'emendamento che hanno messo al centro anche questo tema, dando al Ministro che andrà ad aprire quella trattativa gli strumenti per cercare di dare un margine maggiore alla soluzione di un problema che certamente dovrà vedere nel piano industriale di quell'impresa la risposta più definita e certa; tuttavia, sicuramente avere la disponibilità di sei mesi di cassa integrazione in deroga dà una garanzia, soprattutto ai dipendenti che quel lavoro non vogliono perderlo, di avere gli strumenti per continuare a sopravvivere essendo colpiti

Da ultimo abbiamo affrontato un tema molto importante che riguarda il sisma dell'Aquila del 2009.

che da parte del commissario dell'Unione europea c'è stata un'apertura, una disponibilità, a risolvere questo problema insieme al Governo,

la presentazione delle osservazioni e delle comunicazioni da parte delle imprese rispetto alla procedura che era in scadenza a luglio. Tale termine è stato prorogato proprio per dar tempo al Governo

sia umano che materiale. Quindi abbiamo bisogno, con l'impegno forte del Governo, mostrato anche in Commissione, di risolvere questo problema e dare più certezze a quelle imprese. a quelle imprese. Ribadisco il ringraziamento a tutti coloro che hanno dato un contributo al lavoro della Commissione speciale, che ha lavorato davvero in tempi molto stretti ma con grandissima capacità e competenza.

I subemendamenti agli emendamenti approvati dalla Commissione dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi. Rinvio

in merito ai ritardi accumulati ormai da anni nell'erogazione dei contributi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014‑2020. Si tratta dei contributi destinati all'agricoltura e alla zootecnia, settori di rilevante importanza, soprattutto per una Regione a forte vocazione agricola come la Sicilia, penso anche alla Sardegna e a gran parte del Meridione d'Italia, in cui queste attività possono rappresentare un volano per l'economia locale e una ritrovata fonte di reddito e occupazione anche per i nostri giovani. Ogni anno gli imprenditori rurali si affannano, scontrandosi con una burocrazia soverchiante per rispettare le scadenze previste dal PSR e avere così la possibilità di accedere ai finanziamenti, riponendo in essi grandi speranze, ma a distanza di anni la liquidità è raramente disponibile e le aziende agricole e zootecniche si trovano costrette, ancora una volta, ad attendere e soffrire. Colleghi, non è più concepibile che lo sviluppo rurale del nostro Paese sia ostacolato da procedure fortemente burocratizzate, ereditate da una classe politica fallimentare. *(Applausi dal Ci sono circa 4.600 giovani che hanno presentato la richiesta di insediamento, ormai quasi un anno fa, e ancora non sanno se potranno o no avviare la propria azienda in Sicilia. Ci sono centinaia di imprese nel settore agrozootecnico in attesa di ricevere il pagamento del bando delle coltivazioni biologiche del 2015, del 2016 e del 2017; pagamenti bloccati da tre anni a causa di anomalie generate da un sistema informatico che sta costringendo agricoltori e allevatori ad indebitarsi per sopravvivere, vedendo le loro aziende andare al collasso. A questi lavoratori do la mia piena solidarietà. Rivolgendo ad essi il mio primo intervento in Assemblea, mi impegno sin da subito a farmi carico delle loro istanze, sollecitando i soggetti responsabili, *in primis* Agea, per trovare, unitamente all'autorità di Governo, una soluzione a questa grave problematica che ostacola lo svolgimento delle attività produttive rurali e lo sviluppo del territorio e di grandi aree del nostro Paese.